Senatori, il prossimo 11 agosto sarà il centesimo anniversario della promulgazione della legge che ha disposto la traslazione all'Altare della Patria della salma del Milite ignoto: un atto solenne voluto dal Parlamento per onorare la memoria dei 651.000 soldati italiani caduti durante la Prima guerra mondiale. Il loro sacrificio è testimonianza di alcune delle pagine più drammatiche della nostra storia: pagine di coraggio, pagine di eroismo e altruismo, di cui sono stati protagonisti i nostri soldati, così come delle loro umane paure, delle angosce e delle frustrazioni che nelle trincee di confine accompagnavano lo scoppio di ogni colpo di artiglieria. Pagine scritte con il sangue di tanti giovani che hanno affrontato gli orrori della guerra e con il dolore di genitori, mogli e figli che non li hanno visti tornare a casa, e a cui troppo spesso è stata perfino negata l'intima pietà di una tomba o di una lapide su cui piangere o deporre un fiore. Nel tempo, le spoglie di quel giovane milite senza nome sono diventate il simbolo del grande cuore di tutti gli italiani in divisa, che hanno perso la vita in guerra o in missione ovunque nel mondo; donne e uomini di ogni generazione che hanno difeso con orgoglio, incrollabile senso del dovere e instancabile dedizione, la Patria e i suoi valori; valori che oggi sono le fondamenta di una Nazione libera e dialogante. Un Paese che crede fermamente nella pace come bene comune da proteggere contro ogni forma di violenza o di prevaricazione; un Paese che non dimentica e che, in questo solenne centesimo anniversario, onora i suoi martiri con iniziative meritorie e di valore, come l'idea di riconoscere la cittadinanza onoraria al milite ignoto da parte di tutti i Comuni d'Italia, come il Treno della memoria, che il prossimo 28 ottobre partirà da Aquileia per giungere a Roma il 4 novembre, unendo ancora una volta il Paese in un nuovo viaggio simbolico, sulle orme di quello che un secolo fa portò le spoglie del milite ignoto fino all'Altare della Patria. Soprattutto un Paese che racconta, spiega, tramanda la propria storia alle generazioni di oggi e a quelle di domani, perché si facciano anch'esse messaggere di una memoria che è parte della loro identità culturale, oltre che una guida preziosa per costruire un futuro migliore, perché comprendano davvero l'inestimabile ricchezza di un patrimonio di principi, tutele e garanzie individuali e collettive che è frutto anche di grandi sofferenze e sacrifici di vite umane. Vi ringrazio

ringrazio anche per la cortesia istituzionale che ha voluto usarmi. Intervengo per richiamare l'attenzione di quest'Assemblea e, attraverso di essa, del discorso pubblico della nostra Nazione sul disastro che ha colpito la Regione Abruzzo: una vera e propria strage di alberi che domenica abbiamo purtroppo patito come comunità regionale, a causa di una condotta scellerata di coloro i quali hanno voluto distruggere attraverso il fuoco un patrimonio irripetibile coincidente con il creato. un creato che ci fa pensare, in termini di sentimento, di avvertimento delle coscienze, a quello che lei ha richiamato prima a proposito dell'opera estrema garantita dal Milite ignoto, perché la Patria che evoca il suolo sotto il quale sono sepolti i nostri avi è fatta anche del paesaggio, del creato, di quanto consente memoria individuale e collettiva. In Abruzzo abbiamo perso qualcosa come 100.000 alberi. Un sacerdote di grande credibilità, monsignor Iannucci di Pescara, ha insegnato a numerose generazioni che gli alberi sono i cittadini che avremmo voluto avere in più.

Trabocchi. Intervenire in Senato in questo momento serve a richiamare l'attenzione delle istituzioni. Il codice di protezione civile del 2020 prevede che davanti a questi disastri si attivino le procedure per il riconoscimento dell'emergenza nazionale.

ci fosse solo l'intervento degli organi statuali governativi, non ripristineremmo il valore del Paese saggio che è evocato dal paesaggio. C'è bisogno anche di fare di più ad opera della cittadinanza, ad opera di coloro i quali hanno molto, anche sul piano della ricchezza. Infatti ci vorranno almeno quindici anni per ripristinare quei 100.000 alberi per le giovani generazioni che vorranno rivendicare il diritto alla veduta della bellezza. bellezza. Serviranno norme per scoraggiare questi delinquenti che attraverso il fuoco hanno distrutto il Creato; serviranno sanzioni, risorse per fare in modo che i progetti di carattere ambientale dispongano anche di colonnine che distribuiscono acqua, estintori su misura del rischio, attraverso il principio di precauzione. Il messaggio ulteriore che vorrei mandare attraverso questo intervento è che dobbiamo fare in modo che le vicende vengano evitate a monte e non a valle, perché intervenire a valle richiede risorse in più, richiede ed impone una perdita di diritti delle giovani generazioni. Signor Presidente, vorrei tanto che la cura e la premura dei Ministeri competenti mettessero in evidenza come la provvista finanziaria deve essere su misura dei valori che abbiamo nelle terre alte delle nostre Regioni. La ringrazio per avermi consentito

dalla pineta D'Avalos, denominata dannunziana in quanto il Vate ebbe a comporre una a comporre una poesia, «La pioggia nel pineto», che evocava esattamente quella pineta. È proprio questo il problema: l'incendio è scoppiato di fatto in città ed è stato forse questo

ai quali ovviamente esprimiamo vicinanza, perché perdere patrimonio boschivo, perdere foreste significa perdere un pezzo della nostra vita e della nostra storia. Pescara però all'interno della città ha non solo un parco, non solo un polmone verde, ma un pezzo della propria storia. Per i pescaresi aver perso più di un terzo del patrimonio forestale di un parco, che divenne di fatto più di dieci anni fa una riserva naturale, ha significato perdere un pezzo di storia. Esprimo pertanto un senso di affetto e di solidarietà - mi auguro di poter parlare anche a nome di tutto il Gruppo - nei confronti del sindaco della città di Pescara, Carlo Masci, che addirittura ha pianto dinanzi alle telecamere quando lo hanno intervistato, perché sentiva su di sé la drammatica situazione del patrimonio forestale e storico di una città che andava in fumo, un fumo che addirittura ha lambito abitazioni civili, ha costretto anche molte suore ad abbandonare la propria sede per essere alloggiate presso un albergo della città. Anch'io mi permetto di dire che in situazioni come queste bisogna sensibilizzare tutto il Parlamento affinché si adottino

una notizia nei telegiornali di tutta Italia, ma che può essere un'occasione di vicinanza per gli amministratori locali della città di Pescara e dell'intera Regione Abruzzo. *(Applausi)*.

Signor Presidente, desidero associarmi anch'io alle parole dei senatori D'Alfonso e Pagano per esprimere il mio sconcerto, che deve essere quello di tutti noi, di fronte a questa tragedia che ferisce la città di Pescara. Sono luoghi - quelli che sono stati così ferocemente colpiti e devastati dalle fiamme - particolarmente cari a chi vi parla perché, fra l'altro, nell'immediata prossimità dell'università per tanti per tanti anni ho avuto l'onore di condurre la mia carriera: un polmone verde per la città, a ridosso delle abitazioni e degli stabilimenti balneari. È emersa ancora una volta con una tragica evidenza la fragilità di un territorio meraviglioso, ma esposto troppo spesso alla furia delle intemperie. Questo deve naturalmente suscitare in tutti noi una riflessione: in questo caso è stata la siccità, in altri casi sono state le bombe d'acqua, la grandine, a mettere in seria difficoltà la cittadinanza di Pescara e i suoi amministratori, cui va tutta la mia la mia solidarietà, il mio affetto e la mia vicinanza in questo momento, nonché l'assicurazione - per quello che possiamo nel nostro ruolo di parlamentari del territorio - che tutto sarà fatto per cercare di rimediare agli esiti di questa terribile catastrofe. Ringrazio lei, Presidente, e i colleghi che sono intervenuti per averci consentito di attirare l'attenzione su questo tremendo episodio. *(Applausi)*.

il mio intervento arriva in coda a quello dei colleghi abruzzesi delle altre forze politiche che hanno già ricordato il dramma che in questo momento sta vivendo vivendo l'Abruzzo. E nel ricordare l'Abruzzo non possiamo dimenticare le altre zone del Paese colpite in questi giorni da incendi devastanti, a cominciare dalla Sardegna. Non starò qui a ripetere le cose già dette sui danni, sui rischi che la stessa popolazione intorno a questi incendi e all'interno delle zone degli incendi ha corso e sta correndo. Mi lasci dire una cosa, Presidente, per ricordare anzitutto a me stesso e a tutti che quando si parla di incendi spesso si dimentica di parlare di prevenzione. È a tutti chiaro, per le notizie che stanno arrivando perlomeno dall'Abruzzo, che tali incendi sono frutto di mani dolose che appiccano sistematicamente il fuoco

Voglio ricordare che in Abruzzo, nel mese di luglio, era arrivato l'allarme dei Vigili del fuoco che si lamentavano per il taglio dei fondi antincendio da parte della Regione. Non voglio qui fare polemiche, ma quello che è successo ha dimostrato che l'allarme dei Vigili del fuoco era giustificato e se ne è vista la giustificazione proprio davanti alle dimensioni devastanti dei roghi. Per questo ricordo a tutti noi che, piuttosto che continuare ogni anno a lamentare questi episodi, potremmo più concretamente cercare - anche all'interno del Senato - di avviare un'iniziativa, un'indagine conoscitiva per tentare di capire la dimensione del fenomeno e soprattutto tutti i mezzi che servono e che mancano a quella politica di prevenzione che tutto il Paese si aspetta. Grazie, Presidente.

popolazioni che vivono oggi il dramma degli incendi. Non è solo l'Abruzzo, che già basterebbe ad alzare un campanello d'allarme rispetto, da una parte, ai cambiamenti climatici e, dall'altra, alla stupidità umana di chi appicca fuoco in località così di pregio, come è accaduto a

di prevenzione in un contesto parlamentare quando è stato il Parlamento nella legislatura scorsa a privarsi dell'unico Corpo che in Italia faceva prevenzione e, cioè, il Corpo forestale dello Stato. Cerchiamo di far ritornare il discorso in un alveo un po' più di coerenza e, in qualche maniera, di onestà intellettuale. Quel Corpo non faceva solo repressione, che in tanti casi è dovuta, ma aveva anche - lo dico da sindaco - una grandissima funzione di prevenzione, di assistenza, di collaborazione e di coordinamento assieme alle forze e agli enti istituzionali come i Comuni, le Province e le Regioni.

un progetto di legge presentato alla Camera da Fratelli d'Italia, a mia prima firma, e un disegno di legge al Senato a prima firma della collega Rauti, che potrebbero recuperare

vi è una situazione di grave emergenza. Lo dico anche al presidente D'Alfonso, che, magari, ci può essere d'aiuto per capire come intervenire.

questo serve. Tra poco discuteremo della cybersicurezza, ma abbiamo un problema di sicurezza ambientale e di prevenzione. Abbiamo chiesto varie volte di poter utilizzare i droni e di fare un investimento della Protezione civile e dello Stato in modo da poter sorvegliare

reclutamento abbiamo presentato alcuni emendamenti che riguardano proprio il Corpo forestale, che ovviamente sono stati dichiarati improponibili, ma l'abbiamo fatto per sollevare la questione e chiedere - vedo il collega Toninelli, che ha fatto la stessa richiesta

di riuscire a trovare delle soluzioni per porre rimedio a quello che è stato un errore gravissimo. Non dimentichiamolo, evitiamo

mia personale e penso di tutta l'Assemblea, alle popolazioni che sono state colpite. Mi riferisco non soltanto agli incendi che hanno devastato l'Abruzzo, ma anche a quelli che hanno devastato

ha rivelato i problemi del dissesto idrogeologico. Siamo pertanto in presenza di un'Italia bella, ma molto, molto fragile. finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha ridefinito il calendario della settimana corrente. Nella seduta odierna si discuterà, fino alla sua conclusione, il decreto-legge in materia di cybersicurezza. A tal fine la seduta non prevede orario di chiusura. L'ordine del giorno della seduta di domani, con inizio alle ore 11, prevede la discussione congiunta del rendiconto 2020 e dell'assestamento 2021, per le cui votazioni finali è richiesta la presenza del numero legale. Saranno inoltre rese le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge di delega al Governo in materia di spettacolo, collegato alla manovra di finanza pubblica. La seduta verrà quindi sospesa fino alle ore 16 e riprenderà con la discussione delle risoluzioni approvate dalle Commissioni riunite affari esteri e difesa sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi per complessive tre ore, comprensive delle dichiarazioni di voto, fatti salvi i tempi dei relatori e del Governo. Giovedì 5 agosto sarà discusso il decreto-legge sulla salvaguardia di Venezia e la tutela del lavoro. Il *question time* già previsto per le ore 15 di giovedì non avrà luogo. I lavori delle Commissioni riprenderanno dalla settimana del 30 agosto, ferma restando l'autorizzazione a convocarsi in qualunque momento, anche in data antecedente, in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 7 settembre, alle ore 16,30, con comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori, che sarà definito dalla Conferenza dei Capigruppo convocata nella stessa giornata di martedì 7 settembre, alle ore 15. Ricordo che giovedì 5 agosto, alle ore 8,30, sarà convocata la Commissione monocamerale d'inchiesta sul gioco d'azzardo, per la propria costituzione.

del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in tema di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La relatrice, senatrice Mantovani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in tema di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ricordo preliminarmente che la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e rappresenta uno dei sette investimenti della digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione", compresa nella missione 1 "Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo". Il testo del decreto-legge, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, si compone di 19 articoli. Gli articoli da 1 a 4 definiscono il sistema nazionale di sicurezza cibernetica, che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri. Nello specifico, l'articolo 1 reca alcune definizioni utilizzate nel decreto-legge. L'articolo 2 attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, l'adozione della relativa strategia nazionale, nonché la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale,

L'articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni che non sono attribuite a lui in via esclusiva. L'Autorità delegata è tenuta a informare costantemente il Presidente del Consiglio, il quale, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare a sé l'esercizio di tutte o di alcune funzioni. L'Autorità delegata, in relazione alle funzioni esercitate, ai sensi del presente decreto-legge, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale, di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 22 del 2021. L'articolo 4 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti: proporre al Presidente del Consiglio gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale; esercitare l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza; promuovere l'adozione di iniziative per favorire la collaborazione a livello nazionale e internazionale tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza; esprimere il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto dall'autorità delegata e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Possono partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri e altre autorità civili e militari, di cui di volta in volta si ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare. Infine, sono trasferite al CIC le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal decreto-legge n. 105 del 2019 (cosiddetto decreto-legge perimetro) e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste all'articolo 5 del medesimo decreto-legge in tema di disattivazione di apparati o prodotti in caso di rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale, connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici. Seguono una serie di disposizioni che riguardano l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, organo strumentale all'esercizio delle competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio e all'autorità delegata. L'articolo 5 ne prevede l'istituzione, dotandola di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal decreto in esame. In particolare, il decreto-legge prevede l'adozione dei seguenti regolamenti: regolamento di organizzazione e funzionamento; regolamento di contabilità; regolamento sulle procedure per la stipula di contratti di appalti, di lavori e di forniture per le attività finalizzate alla sicurezza; regolamento del personale. L'articolo 6 disciplina l'organizzazione dell'Agenzia, al cui vertice figura il direttore generale, che è il legale rappresentante dell'Agenzia, nonché il diretto referente del Presidente del Consiglio e dell'autorità delegata. L'articolo 7 definisce le numerose funzioni dell'Agenzia, riconosciuta come autorità nazionale per la cybersicurezza, come autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nonché come autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza. Ulteriori disposizioni riferite all'Agenzia si rinvengono nell'articolo 11, relativo a risorse finanziarie e autonomia contabile; nell'articolo 12, che disciplina il personale, e nell'articolo 14, con riferimento alle relazioni annuali che il Presidente del Consiglio è tenuto a trasmettere al Parlamento e al Copasir sull'attività dell'Agenzia. Gli articoli 8 e 9 riguardano la costituzione, presso l'Agenzia, di un nucleo per la cybersicurezza per gli aspetti relativi alla prevenzione e alla preparazione a eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. L'articolo 10 riguarda la gestione delle crisi che coinvolgano aspetti della cybersicurezza. L'articolo 13 ha per oggetto la trattazione dei dati personali per finalità di sicurezza nazionale e cibernetica. L'articolo 15 detta una serie di novelle al decreto legislativo n. 65 del 2018, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2016/1148, cosiddetta direttiva Network and Information Security al fine di armonizzarlo con l'impianto normativo proprio del decreto-legge in esame. L'articolo 16 novella al medesimo scopo altri atti normativi. L'articolo 17 reca disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 18 contiene disposizioni finanziarie. L'articolo 19 dispone in merito all'entrata in vigore. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà. Presidente, membri del Governo, colleghi, l'asciutta relazione che abbiamo appena ascoltato nelle parole della relatrice dà sicuramente un'idea dell'architettura di un sistema, ma forse non riesce a darci fino in fondo la dimensione profonda che i problemi di *cybersecurity* hanno sotto una serie di aspetti che ci toccano molto da vicino. Nel caso concreto mi piace soffermarmi sull'impatto che tali aspetti hanno in tema di salute. Voi sapete - è parte integrante del Piano che la transizione digitale rappresenta il presupposto per consentire alle organizzazioni che compongono il Sistema sanitario nazionale di raggiungere gli obiettivi che sono stati messi a fuoco proprio nella grande operazione di modernizzazione del nostro Paese,

per aprirla ad abbracciare le infinite misure che possono riguardare una sanità più attiva sui territori. La transizione digitale assume perciò una rilevanza strategica e trasversale rispetto a tutti gli altri temi trattati. Per tale motivo occorre semplificare l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali, anche ridisegnando un modello di Sistema sanitario nazionale che sappia accompagnare il paziente fin dall'inizio della fruizione dei servizi, includendo la continuità ospedale-territorio, l'integrazione, la collaborazione sociosanitaria, lo sviluppo dell'assistenza domiciliare, grazie alla definizione di adeguati percorsi diagnostico-terapeutici. Ma nulla di tutto ciò potrebbe essere fatto senza una forte, chiara, esplicita e - mi si passi il termine - rivoluzionaria transizione tecnologica, che consegni al sistema digitale la gestione di dati di una delicatezza infinita, come sono tutti i dati che riguardano la nostra salute e, in un certo senso, la nostra identità personale. È la grande rivoluzione che la tecnologia farà attraverso la transizione digitale, di cui - attenzione - si assume in prima persona la responsabilità il Presidente del Consiglio. Il tema della *cybersecurity* ha nel Presidente del Consiglio il suo punto di riferimento e noi ci auguriamo che - costi quello che costi - la transizione si faccia a garanzia della salute, a garanzia dei dati e della *privacy* di ognuno di noi, a garanzia dell'efficacia e dell'efficienza. Proprio per questo nella 12a Commissione, discutendo oggi

l'Assemblea: nella cabina di regia, tra le tante autorevoli persone chiamate a farne parte, ci sia anche il Ministero della salute.

Credo che questo possa essere un momento molto positivo per modificare in meglio il Sistema sanitario nazionale e generare quei piani nazionali che finora

Signor Presidente, il recentissimo attacco *hacker* al sistema informatico della Regione Lazio ci ha fatto comprendere, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la minaccia cibernetica è in realtà concreta e prossima alla vita dei cittadini comuni. I *malware*, sempre più sofisticati, non solo offendono gli interessi strategici del Paese, ma possono anche colpire direttamente le persone, sottraendo loro risorse economiche, accesso alle fonti energetiche, ai trasporti e alle cure. questo attacco si sarebbe trattato di un *ramsonware* con finalità estorsive, che ha creato un ritardo nel funzionamento del sistema regionale di vaccinazione, che opera nell'ambito dell'efficiente dell'efficiente coordinamento nazionale affidato alla professionalità del grande generale Figliuolo, e potrebbe essere stato la causa di altre infezioni che si sarebbero potute naturalmente evitare. Lo stesso tipo di attacco ha recentemente paralizzato il sistema sanitario irlandese e il grande oleodotto americano. Anche durante le guerre, le istituzioni sanitarie del nemico sono protette da convenzioni internazionali; gli attacchi informatici, invece, non hanno regole e i loro scopi spesso non sono facilmente decifrabili, come l'identità dei loro autori. Non possiamo dunque che giudicare opportuna e necessaria l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che colma un vuoto ormai anacronistico tra gli strumenti per la difesa degli interessi e degli *asset* nazionali. La delicata fase della transizione digitale della pubblica amministrazione deve essere protetta e guidata dagli esperti dell'Agenzia, anche per evitare che si perpetui che si perpetui l'assurda situazione che i sistemi informatici delle istituzioni siano notevolmente più fragili e arretrati rispetto ai sistemi detenuti dai privati. sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni contengono i dati più riservati dei cittadini e dovrebbero essere difesi dalle incursioni criminali, con la stessa cura riservata ai servizi segreti vitali dello Stato. La sicurezza dei dati dei cittadini diventerà ancor più cogente dal momento che verrà creato il fascicolo sanitario elettronico omogeneo a livello nazionale, che diventerà il singolo punto di accesso, per cittadini e residenti, alla propria storia clinica e ai servizi offerti dal Servizio sanitario nazionale. Altro aspetto della trasformazione digitale della pubblica amministrazione, prescritta dal PNRR, sarà la migrazione delle amministrazioni sul *cloud* e l'interoperabilità dei sistemi informatici, accentramento telematico che dovrà avvenire in un ambiente rigorosamente presidiato. Auspico che l'Agenzia possa essere una struttura agile e reattiva e non posso che apprezzare il fatto che essa risponderà direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento. Ma il rafforzamento della cybersicurezza del comparto pubblico potrebbe essere inefficiente se non si provvederà a una robusta campagna di informazioni al largo pubblico sui temi della sicurezza informatica. Colleghi, noi tutti sappiamo che anche un solo *personal computer* infettato può essere la base di partenza di attacchi informatici devastanti. L'educazione alla sicurezza informatica dovrebbe essere materia di insegnamento, come lo è la sicurezza stradale. L'Agenzia sarà il centro nazionale di coordinamento che si rapporterà con gli omologhi organismi internazionali, un presidio importante per la protezione dei nostri cittadini che avvicinerà l'Italia ai più alti *standard* di sicurezza. *(Applausi)*. Grazie, Presidente. del Governo, come ha detto bene il relatore, la *cybersecurity* è il pilastro fondamentale dell'economia digitale ed è per questo che dobbiamo intendere l'Agenzia

definendo le *partnership* tra pubblico e privato. A tal proposito, apro una parentesi. Una serie di gare d'appalto è stata aggiudicata a fornitori privati e nei capitolati non si è prestata alcuna attenzione ai temi della *cybersicurezza.* Tenete presente che una parte significativa di di manutenzione applicativa e ai sistemi viene fatta proprio da aziende private

auspicabile una forte cooperazione internazionale tra le Agenzie di *intelligence* perché è fondamentale conoscere il nemico. Il nemico del terzo millennio

ospedali, la comunicazione e tutto ciò che vive e funziona attraverso le connessioni. *(Applausi)*. Pensate addirittura che oggi delle mani esperte potrebbero bloccare un'auto di ultima generazione

e, se vogliamo, anche inconsapevole - tutto quello che possediamo. E ciò avviene perché non abbiamo mai investito sulla formazione generalizzata e diffusa

lo vediamo quotidianamente - e la sicurezza dei nostri sistemi informatici assume una centralità assoluta. Nulla è più come prima. Come ricordava la collega Tiraboschi, abituati a conflitti internazionali di stampo bellico, con l'utilizzo magari di carri armati, di razzi, di aerei, ma oggi siamo di fronte a uno scenario completamente diverso, che ci deve far riflettere

Dobbiamo reagire e credo che la risposta che stiamo dando quest'oggi sia adeguata, ma dobbiamo sicuramente fare di più. Dobbiamo imparare a proteggere i nostri confini,

dare un monito, soprattutto alla politica, facendo attenzione anche alla classe dirigente che sarà chiamata a guidare il Paese: già sono stati 300 gli assunti, ma abbiamo necessità di avere personale altamente qualificato.

si trovò di fronte a una situazione gravissima: se è vero che aveva radar e mezzi bellici molto importanti, è altrettanto vero che non riusciva a decodificare il codice enigma che veniva utilizzato dall'Asse.

così da decodificare il codice enigma. A farlo furono linguisti, giocatori di scacchi, matematici, scienziati, persone di altissimo livello. Noi abbiamo la necessità di ricercare

Dobbiamo rispondere con forza; non basta probabilmente il codice penale, con l'articolo 615-*ter* e, soprattutto, con la previsione

nell'ottica della progettazione del futuro, una delle sfide più grandi e più complesse che dovranno affrontare tutte le società del mondo. Due sono i punti di partenza da analizzare: il primo riguarda il rischio e sostanzialmente la vulnerabilità a cui è esposto il sistema informatico; il secondo riguarda il fatto che il dominio digitale sarà sempre uno dei fattori

gli esempi che si sono succeduti nel mondo negli ultimi anni, per non parlare della vicenda che ha riguardato la Regione Lazio recentemente. Gli attacchi informatici determinano dei costi per il sistema, costi legali, costi normativi e costi informatici, e c'è bisogno di dare delle risposte per ridurre tali costi e i rischi per i nostri cittadini. è stato fondamentale far crescere una radicata cultura della cybersicurezza, perché sono esposti ai rischi le pubbliche amministrazioni da un lato, ma anche il tessuto economico privato dall'altro. Spesso, il tessuto economico, soprattutto quello delle piccole e medie imprese, è molto esposto, perché i sistemi di sicurezza delle stesse sono deboli e le imprese non hanno le risorse sufficienti per far fronte

sono stati un rafforzamento delle Commissioni, un rafforzamento del ruolo del Copasir e un'azione di monitoraggio del Parlamento che dovrà essere svolta anche in futuro per quanto riguarda le iniziative che deve mettere in campo

amministrazione ha un *server* piuttosto esposto da questo punto di vista. Ben venga quindi questo tipo di iniziativa. L'obiettivo dovrà essere una connettività sempre maggiore e diffusa ovunque, che è il carattere fondamentale delle società moderne. Dobbiamo guardare avanti: la rete e l'informatizzazione nuove prospettive di crescita sul piano occupazionale e su quello dei servizi. Dobbiamo proteggere le reti e l'informatizzazione. Non dobbiamo girarci dall'altra parte, ma anzi dobbiamo sostenere con convinzione il progresso. Noi riformisti accettiamo questa sfida, non ci chiudiamo a riccio, non abbiamo lo sguardo rivolto al passato, ma anzi guardiamo al futuro crediamo che la società vada cambiata e resa più sicura. In questo senso, l'impegno che il Governo ha manifestato con il provvedimento in esame viene fortemente sostenuto dal Parlamento in maniera

l'analisi dello stato di avanzamento dell'Agenzia e del suo funzionamento, che è l'aspetto cruciale del decreto-legge in conversione che ci apprestiamo ad approvare. la questione della cybersicurezza e della sicurezza informatica è estremamente importante. Sempre più affidiamo i nostri dati di ogni tipo alla Rete, a supporti informatici; indubbiamente ciò velocizza una serie di processi e consente di realizzare una serie di comodità e di economie

ci espone a particolari pericoli e ciò vale per tantissimi ambiti, dalla sicurezza militare, alla sicurezza governativa, a quella delle strutture del Governo, dei dati sanitari, dei dati bancari. È una serie difficile da completare, perché oramai tutti i nostri settori si affidano a questo supporto, a questa tecnologia. La sicurezza in questo campo è dunque fondamentale, come è già stato detto. Altri Paesi sono molto più avanti di noi, hanno delle strutture che già lavorano da anni, con grande grande supporto di mezzi e di personale. Noi siamo indietro. Il Governo precedente ha fatto il possibile per farci rimanere indietro con degli stravaganti progetti di affidare la gestione

perché nelle università più serie e accreditate, dove l'ingegneria informatica è ai massimi livelli, le esercitazioni principali per quanto riguarda la sicurezza, che - come sappiamo benissimo - è fondamentale, vengono fatte nel modo seguente: metà degli studenti lavora come se fosse una banca, un Ministero, un'azienda, una entità che abbia interesse a tutelare i propri dati e a non far entrare estranei; un'altra metà degli studenti fa il lavoro opposto, quello dello *hacker,* del pirata cibernetico. Dico questo per

società, l'entità, il Ministero, il reparto militare che riesce a mantenere la propria sicurezza, mentre al secondo c'è il soggetto che non riesce e cioè perde. Bisogna

della quantità, per cui bisogna dotarsi delle strutture, delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie,

È stato inserito questo comma, nel quale si dice che ai componenti del nucleo non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Questa è una bellissima, virtuosa, direi affermazione, ma ho qualche dubbio che sia possibile attirare le competenze necessarie a queste condizioni: zero soldi, zero compensi, zero rimborsi spese.

avere un approccio assolutamente strutturale, perché qui non c'è differenza tra militare e non militare, tra un settore e l'altro, fra l'interno e l'estero: globale, la minaccia dunque è globale, può arrivare da qualunque parte del pianeta, naturalmente può anche arrivare dall'interno del nostro Paese e la vittima può essere chiunque. Non c'è neanche una distinzione dal punto di vista della vulnerabilità e della strategicità strategicità delle possibili conseguenze di un attacco che subiamo e che tale attacco abbia successo, perché non c'è differenza tra pubblica amministrazione e privati, perché non c'è differenza tra colpire

viene un po' tenuta da parte. Questo è un tema di interesse nazionale, che interessa tutti, non si può escludere nessuno, non si possono includere nel comitato ministeriale alcuni Ministeri, magari perché oggi sono occupati da esponenti di certe forze politiche o di certe correnti culturali, e tenerne fuori C'è un gran lavoro da fare, questo è un primo passo ma la questione della cybersicurezza deve essere trattata con grande serietà e con la coscienza che ci coinvolge tutti, che c'è bisogno della collaborazione di tutti, delle menti e delle idee migliori. Abbiamo presentato i nostri emendamenti e ordini del giorno per dare un contributo, bisogna andare avanti e molto su questa strada.

Signor Presidente, che ci volesse un'Agenzia per la cybersicurezza l'avevamo detto più volte;

si è ripreso un cammino rispetto a questo tema e proprio in questi giorni - nella vita serve anche la fatalità

sarei curiosissimo di sapere nel dettaglio quanti colleghi hanno letto tutti gli articoli del decreto-legge sulla cybersicurezza. seppur siamo totalmente d'accordo sull'istituzione dell'Agenzia, vorrei chiedere a tutti

Mi piacerebbe sapere se tutti hanno letto che gli stipendi delle 300 persone che vi lavoreranno sono adeguati alla Banca d'Italia, soggetto di diritto privato, quindi non legato ai tetti. Poi non vi lamentate se gli stipendi sono alti! D'altra parte, è anche giusto che sia così, ci mancherebbe altro. Tuttavia, nella vita serve coraggio: se vogliamo fare questa scelta attiviamo lo *spoil system*, assumiamoci la responsabilità, andiamo a scegliere i migliori.

Mi è stato detto che è un accordo nato così. A me non piace: si parla di funzione pubblica, si parla di uffici pubblici, di sicurezza dello Stato,

è abbastanza singolare. L'ultima questione sulla quale voglio spendere il tempo che mi resta è il ruolo del Parlamento. C'è un articolo all'interno della norma che dice che il Copasir può convocare il direttore generale dell'Agenzia: ma questa è una grande fortuna! Meno male che ce lo dice la legge, meno male. Signori, in queste settimane, in questi mesi, il Parlamento sta perdendo ogni giorno ruolo, funzione, qualità. Stiamo attenti: non vorrei che prima o poi nascesse un'agenzia parlamentare che ci sostituisse tutti.

Signor Presidente, userò molto meno del tempo che mi è stato assegnato; sarò molto breve anche perché - è giusto dirlo - questo provvedimento ci arriva dalla Camera dei deputati e, come spesso accade ultimamente, con scarso margine di manovra; quindi, anche l'esame in Commissione è stato abbastanza rapido. È giusto ricordarlo e sottolinearlo tutte le volte perché credo che ribadire ogni volta, indipendentemente dal nostro ruolo di maggioranza o di opposizione, la difesa della centralità del Parlamento sia per noi prima di tutto un dovere.

perché si tratta di un provvedimento fondamentale anche per attuare i nostri impegni legati al PNRR. È un provvedimento importante per la vera emergenza che - permettetemi - non è esagerato paragonare alla situazione legata al covid. Non si vede, ma da alcuni anni è in corso una vera e propria guerra che non si combatte più sui campi di battaglia, ma lungo le linee di comunicazione informatica. Forse definirla una terza guerra mondiale è esagerato, però è davvero una situazione difficilmente quantificabile e valutabile dai più. È importante che il Parlamento assuma consapevolezza di ciò che è al giorno d'oggi la cybersicurezza e che si agisca anche perché l'utilizzo di tecnologie informatiche, come è ovvio che sia, aumenta in modo esponenziale di anno in anno. Nell'ultimo anno abbiamo visto quanto tutto ciò che è legato allo *smart* *working* ci ha portato ad aumentare la diffusione di dati che si muovono lungo le linee telematiche anche in settori che prima ne erano toccati solo marginalmente e, quindi, la cybersicurezza è un tema centrale della nostra politica. Anche gli attacchi aumentano in modo esponenziale ed è un settore dove l'evoluzione di questi attacchi è sempre crescente. Volendo fare un paragone, visto che siamo in giornate di eventi sportivi poiché sono in corso i giochi olimpici, direi che dobbiamo agire come l'antidoping che deve seguire il *doping* in continua evoluzione. C'è un *doping* informatico che ogni giorno si evolve e aumenta le proprie capacità e noi dobbiamo inseguire, essere aggiornati e permettere a tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte di essere sempre pronte a rispondere a questi attacchi, che mutano giorno dopo giorno. Non è un tema facile; è un tema delicato, lo sappiamo. Bisogna agire con decisione, ma anche con cautela

È importante che il Parlamento ci sia, venga coinvolto e che in questo modo ci sia anche la possibilità di tenere un rapporto diretto con i cittadini elettori.

*hacker*. Scopriremo i dettagli più avanti, ma possiamo dire che è un attacco informatico fatto per fare male e che ha mostrato le debolezze del nostro sistema, non solo perché vengono trafugati i dati, cosa che già di per sé è grave, ma perché viene compromesso e messo in pericolo l'intervento sulla salute pubblica ed è inutile che vi ripeta quanto ciò sia importante in questo periodo. periodo. Dobbiamo intervenire al più presto per dare strumenti a tutte le nostre istituzioni per affrontare questa sfida. Lo dico anche se avrei potuto - e avrei avuto gioco facile attaccare la scarsa lungimiranza di quel Presidente di Regione che un anno fa prendeva gli aperitivi sui Navigli. Ce lo ricordiamo,

Avremmo ascoltato il senatore Pellegrini chiedere le dimissioni di Fontana? Avremmo sentito il senatore Toninelli chiedere il commissariamento della Regione Lombardia? Sono lontano dalla realtà? No, avremmo sentito queste frasi; avremmo ascoltato, magari dalla sinistra, accuse alla Regione Lombardia di aver messo in pericolo delle vite.

Dicevo che avrei gioco facile ad andare avanti per tutti i miei dieci minuti e potrebbero accodarsi tutti i colleghi del Gruppo.

di questo è la misura del nostro essere qui, il nostro essere in Parlamento e di essere al Governo con responsabilità.

Presidente, farò una breve replica. Sono sicuramente soddisfatta di sentire da tutte le forze politiche che c'è unità e concordia sulla necessità dell'istituzione di questa Agenzia,

sulla necessità di una formazione più pervasiva, in quanto oggi abbiamo una forte carenza di queste professionalità ed è necessario

Per quanto riguarda l'attenzione alle piccole e medie imprese, è necessario un supporto, che verrà da tale Agenzia, una maggiore interazione tra le necessità di sicurezza delle piccole medie imprese e della pubblica amministrazione. L'Agenzia potrà offrire il supporto necessario a migliorare la sicurezza di tutti. Una piccola precisazione invece per il senatore Malan, per quanto riguarda i compensi che non spettano al nucleo: il nucleo è un organo consultivo composto dal direttore generale dell'Agenzia, dal consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri e da alte cariche, che hanno già i propri emolumenti. emolumenti. Per quanto riguarda il personale dell'Agenzia, è previsto all'articolo 12 un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia.

Governo,

che conseguentemente il testo sia riformulato in modo corretto grammaticalmente: «valutare l'opportunità di prevedere, per imprese operanti in settori strategici e pubblica amministrazione, l'adozione di strumenti

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'assoluta impossibilità di prenotare ogni tipo di visita medica, incluse le vaccinazioni anti-Covid, il sito della Regione irraggiungibile per giorni e i dati di tutti gli utenti in balia di criminali sconosciuti, interessati solo a richiedere chissà quale tipo di riscatto. L'attacco *hacker* di questi giorni al sistema sanitario della Regione Lazio è la dimostrazione plastica di quanto sia urgente definire una politica nazionale di sicurezza cibernetica, anche perché l'esperienza insegna che le incursioni cibernetiche ad un Paese colpiscono frequentemente aspetti nevralgici del Paese stesso (sistemi aeroportuali, banche, turbine elettriche), come pure grandi aziende del settore privato, bloccate nella loro operatività e messe sotto ricatto attraverso estorsioni milionarie. È recente, ad esempio, il caso della manipolazione telematica a danno della più grande catena di supermercati svedese, costretta a chiudere per giorni oltre 800 punti vendita. Oppure l'attacco *hacker* da parte del gruppo russo Revil a migliaia di aziende statunitensi, che ha mandato in *tilt* decine di migliaia di *computer* in tutto il mondo. esempi calzanti, che fanno capire quanto sia necessario che anche il nostro Paese si doti di uno strumento idoneo a proteggere le funzioni essenziali dello Stato da minacce informatiche, alzando il livello di protezione dei dati e dei sistemi di controllo. Ad oggi si stima che le imprese italiane subiscano ogni anno mediamente 7 miliardi di euro di danni a causa di attentati digitali e solo poche settimane fa abbiamo appreso con sgomento dalle parole del ministro Colao che almeno il 95 per cento delle piattaforme di cui si serve la nostra pubblica amministrazione non è in sicurezza. Ecco perché la realizzazione di un'Agenzia per la *cybersecurity* non è più rinviabile. C'è bisogno urgentemente di dotarsi di uno strumento efficace, che difenda i comparti strategici della nostra sicurezza nazionale dai pericoli rappresentati dalla crescente pirateria informatica, così da tutelarci da possibili aggressioni provenienti da altri Paesi o da forze destabilizzanti e antidemocratiche. L'Agenzia per la cybersicurezza deve rispondere a due missioni principali: innanzitutto alla cosiddetta cyber-resilienza, cioè il consolidamento della collaborazione ai fini della sicurezza cibernetica con l'insieme degli operatori strategici che operano nel settore delle telecomunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della difesa, dello spazio e dell'economia, dalla cui integrità dipende il funzionamento del sistema Paese. In secondo luogo, l'Agenzia dovrà fungere da centro di coordinamento nazionale per gli investimenti nella sicurezza cibernetica. In sostanza, possiamo contare su un organismo in grado di connettere aziende piccole e grandi, capace di coinvolgere le università e la ricerca e di potenziare l'industria del settore rendendola impermeabile ad infiltrazioni ostili, anche da parte di Paesi stranieri. L'Agenzia che andiamo ad istituire con il voto odierno evita la sovrapposizione di compiti con il comparto *dell'intelligence*; è collocata sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio, di conseguenza non è soggetta necessariamente a vincoli di segretezza. Diventa un organismo rapido, snello, adeguato alla complessità della sfida, in grado di svolgere una copertura a 360 gradi ed è virtuoso, perché prevede una *partnership* strutturata e continua tra soggetti pubblici e privati, che lavorano assieme nell'ambito di un'autentica strategia nell'ambito di un'autentica strategia nazionale di sicurezza. Inoltre, la creazione di un'Agenzia nazionale avrà effetti positivi anche dal punto di vista economico; proteggendo in maniera efficace il nostro spazio cibernetico, rendiamo l'Italia più attraente anche per investitori nazionali e stranieri. È il caso di dire quindi che la ripartenza dell'Italia passa anche da qui, da un'Agenzia nazionale in grado di mettere in sicurezza il Paese anche sotto il profilo cibernetico. Noi siamo fortemente convinti della necessità di accelerare i processi di digitalizzazione della società e della pubblica amministrazione, allo scopo di modernizzare il Paese; al tempo stesso siamo consapevoli dei forti rischi legati a possibili attacchi informatici alle istituzioni e ai singoli. Per di più la nostra pubblica amministrazione è in procinto di spostare tutti i propri dati su un *cloud* nazionale, vale a dire su uno spazio di stoccaggio digitale che ci espone ad ulteriori, possibili attacchi. Pertanto, la necessità di tutelare il Paese dalla minaccia cibernetica è uno dei *dossier* più delicati, per noi come per ogni moderna democrazia. Si tratta di una questione di sicurezza nazionale e, al tempo stesso, anche di politica estera. Ci troviamo, infatti, in una fase storica nella quale diversi Paesi, dalla Russia alla Cina, mirano ad acquisire un vantaggio geopolitico attraverso la loro supremazia tecnologica. Un tempo la geopolitica aveva un notevole influsso sulla tecnologia, oggi accade il contrario: la capacità di dotarsi di tecnologie innovative attribuisce un vantaggio strategico in termini di esercizio del potere. Basta guardare quale effetto sta avendo sugli equilibri internazionali il predominio cinese del 5G, cioè la nuova rete digitale di quinta generazione di supporto alla telefonia mobile. Questo è il motivo per cui occorre porre un'attenzione particolare al concetto di sovranità tecnologica ed è necessario che ci allineiamo in fretta all'interno dell'Unione europea, così da colmare il ritardo esistente in materia di nuove tecnologie e dotarci di una vera e propria sovranità tecnologica a livello europeo, che ci permetta di tutelare i nostri commerci, la nostra economia i nostri valori e che determini la nostra autonomia strategica, vale a dire la possibilità di intervenire da soli per fronteggiare possibili aggressioni. Gli attacchi cibernetici sono una minaccia potenzialmente letale per ogni sistema democratico, perché rischiano di mettere in ginocchio settori essenziali di un Paese: centrali elettriche, rifornimenti idrici, discariche di rifiuti; in altre parole, tutti i sistemi vitali di un Paese. Per questo serve una visione comune in materia di cyberdifesa a livello nazionale ed europeo: esattamente ciò che cerchiamo di fare con questo decreto-legge, col quale ci adeguiamo agli *standard* europei e ci dotiamo di una sorta di scudo di difesa dalle aggressioni digitali. Contemporaneamente, mandiamo anche un messaggio all'esterno, a quei Paesi dai quali provengono gran parte degli attacchi cibernetici. Diciamo forte e chiaro che l'Italia è fermamente determinata a non lasciarsi mettere sotto scacco. In sostanza, signor Presidente, la tecnologia sta cambiando passo: porta con sé vantaggi, ma anche rischi, ed è necessario che ci attrezziamo di conseguenza, anche e soprattutto in una fase come quella attuale, in cui si realizza una profonda interrelazione tra la nostra quotidianità e l'informatica. Via via stiamo affidando gran parte della nostra stessa esistenza alla tecnologia: abbiamo un'identità digitale con la quale possiamo accedere a tutta una serie di servizi dal nostro pc. Possiamo ormai fare di tutto con il nostro cellulare, tante nostre informazioni delicate e sensibili sono contenute all'interno di sistemi informatici complessi, così che i dati personali di un soggetto sono sempre più appetibili, purtroppo anche per *hacker* e criminali informatici. Questo è il motivo per cui la sicurezza cibernetica e la tutela dei dati non sono più soltanto un concetto astratto, ma riguardano la vita di tutti noi, il nostro quotidiano. La società tutta sta subendo profondi cambiamenti: grandi istituzioni come la scuola, il Servizio sanitario nazionale, la pubblica amministrazione, come pure il mondo economico produttivo, negli ultimi anni stanno ricorrendo sempre più frequentemente al digitale, dallo *smart working* al *green pass*, dalla didattica a distanza alla telemedicina, tutti strumenti di grande utilità, che allo stesso tempo però ci espongono a rischi finora inimmaginabili. Ecco perché c'è bisogno di strumenti di protezione adeguati come l'Agenzia nazionale per la sicurezza cibernetica, come l'Agenzia nazionale per la sicurezza cibernetica, che rappresenta un nuovo tassello di quell'Italia che stiamo costruendo con il Governo Draghi, moderna ed efficiente, che punta all'innovazione e alle nuove tecnologie, ma capace al tempo stesso di tutelare i diritti delle cittadine e dei cittadini, cosicché l'Italia del domani inizi già oggi. *(Applausi)*.

destino: è singolare che oggi affrontiamo un provvedimento sull'architettura nazionale, sulla cybersicurezza e sull'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nazionale la coincidenza vuole che questo accada dopo un attacco *cyber* al Centro elaborazione dati (CED) del Lazio, del Lazio, che ha mandato in tilt la sanità della Regione. Partiamo dalla cronaca per andare oltre: voglio sottolineare che fino al 13 agosto non si potranno prenotare altri vaccini negli *hub* del Lazio, mentre la mannaia del *green pass* del 6 agosto è davanti a noi e si sta per abbattere su tutti quelli che sono in partenza; e non sappiamo se è solo l'inizio. *(Applausi)*. Basta leggere i giornali di oggi: la paura, il silenzio e l'idea che ci sia un ricatto. Insomma, non sappiamo se è solo l'inizio e se questo attacco vuole arrivare ad altro e colpire altri obiettivi più ampi o se è la sanità il vero obiettivo; chi lo sa. chi lo sa. Sicuramente la situazione è seria - non da oggi - ed è necessaria - non da oggi - l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza.

organica sulla *cybersecurity* e a un rafforzamento cibernetico in vari settori (sanitario, produttivo, industriale e della pubblica amministrazione) anche per i singoli cittadini, che sono tutti utenti del cyberspazio. molto prima che nel contesto del PNRR si inserisse il tema della transizione digitale, Fratelli d'Italia chiedeva, con tutti gli strumenti a dell'Agenzia e sottolineava la necessità di reti resilienti. Abbiamo denunciato più volte il ritardo accumulato su questo fronte e la necessità di una garanzia di sicurezza nazionale nazionale finalizzata alla sovranità digitale. È dal settembre 2020 che il Governo ha assunto un impegno che non ha mantenuto. Ci siamo trascinati fin qui con un ritardo anche perché - com'è noto - con la crescita delle reti è aumentato anche il rischio di violazioni e quindi il dominio *cyber* (la cosiddetta quinta dimensione) è diventato la nuova frontiera e la linea di confronto a livello geopolitico. Cari colleghi, non vi sfuggirà che esplorare lo spazio cibernetico significa entrare in un teatro operativo.

(*cyber)*, che decide della sicurezza globale. Non è un caso se nell'ultimo vertice NATO, in cui è stata approvata la nuova *cyber defense policy*, la minaccia cibernetica è stata equiparata ad altre tipologie di attacco sufficienti per attivare il famoso articolo 5 del Trattato, che coinvolge anche gli altri Paesi alleati a intervenire. È evidente a tutti che siamo in un mondo sempre più interconnesso non soltanto a causa della pandemia e che questo aumento determina un'impennata dei rischi di hackeraggio e una minaccia di attacchi *cyber* sempre più sofisticati e con vari obiettivi, come sottrarre dati per fini predatori e rubare la proprietà intellettuale e l'identità, ma anche - attenzione - obiettivi molto più ambiziosi, come per esempio manipolare informazioni, danneggiare infrastrutture e bloccare erogazioni di servizio, per non parlare del proselitismo dei radicali violenti che si fa *online* e dello spionaggio industriale e militare. Questa è la vera trincea. non è bastato quanto contenuto nella relazione annuale dei nostri Servizi, in cui si è sottolineata la criticità nella sicurezza informatica. Sono ormai note la vulnerabilità

perché il tema della sicurezza nazionale non nasce oggi, ma è un'emergenza che si è imposta da tempo. L'Agenzia dedicata era una necessità e un'opportunità

oggi, perché i Governi ci hanno portato fin qui e non ci potete accusare di ostruzionismo. Siamo stati collaborativi e propositivi appena stati accolti più di dieci ordini del giorno di Fratelli d'Italia - però è imperdonabile il ritardo colpevole con il quale nasce l'Agenzia.

ma lo sapevamo già e lo sapevamo bene. Voglio rammentare che la direttiva europea è del 2016 e che nel 2017 l'Italia annunciò dell'Agenzia, che però non ci fu. Voglio sottolineare che nella bozza della legge di bilancio comparve a un certo punto

Questi ritardi sono vostri, sono una responsabilità, perché stiamo parlando di attacchi che possono comportare il collasso di un sistema; stiamo parlando della nuova sfida sistemica

una lezione al vostro ritardo colpevole, non è certo mettere in dubbio la validità, la necessità, l'urgenza e l'importanza di quest'Agenzia. Attenzione, Attenzione, però, perché la sfida è alta e importante e non si risponde a una sfida strategica con un carrozzone politico. Quindi fate l'Agenzia: fatela subito, fatela bene e fatela funzionare. In ogni caso, il ritardo con il quale arriviamo oggi qui è vostro ed è una responsabilità da cui nessuno vi potrà assolvere.

l'hackeraggio dei dati sanitari della Regione Lazio pone questa nostra discussione in una situazione di drammatica e stretta attualità. Lo hanno notato alcuni colleghi e non c'è dubbio, quindi, che il Parlamento stia parlando di qualcosa cui il Paese guarda con estrema attenzione e preoccupazione. Che sia necessario correre sulle decisioni che riguardano la cybersicurezza lo stanno dicendo in molti in questi giorni. Lo ha detto l'Autorità delegata in una recente intervista,

dire una parola di polemica sul Covid-19 o sulle situazioni che lo riguardano: non l'ho fatto mai per scelta; non perché a volte non potesse essere utile farlo, ma non l'ho fatto.

Questa esigenza di correre, signor Presidente, non è che il Parlamento non l'avesse recepita già prima. In Commissione difesa

al Ministero degli interni e al Ministero della ricerca. Abbiamo udito poi anche grandi aziende, perché il problema non riguarda soltanto il settore pubblico. Presidente, un quadro di grande allarme. Nelle audizioni che abbiamo svolto, è stato evidenziato l'aumento esponenziale degli attacchi cyber, ulteriormente incrementati nel periodo Covid, per lo *smart working* e per le situazioni che si stavano creando. sono impressionanti. Il tema legato al rischio dei dati sanitari, che oggi stiamo mettendo in evidenza per quello che riguarda la Regione Lazio, in Commissione difesa era già stato sottolineato dalla dottoressa Nunzia Ciardi, direttrice del servizio della Polizia postale, che ha fatto un'audizione brillantissima, molto interessante.

altamente qualificato, perché stiamo parlando di una materia con un'evoluzione così rapida che, se non stiamo al passo con i tempi, i cosiddetti cattivi diventano molto più forti di noi.

L'Agenzia ha una personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, ed avrà il compito di svolgere il ruolo di Autorità nazionale, come ricordava prima un collega di Forza Italia, attuando una centralizzazione delle funzioni e delle competenze che finora erano distribuite fra enti e Ministeri: questa era la principale fragilità, perché è necessaria una risposta unitaria e le risposte non possono essere frammentate.

Ricordo che dal 1991 ad oggi si sono succeduti Governi di cui hanno fatto parte anche esponenti che oggi sono in Fratelli d'Italia. Lo dico perché, se vogliamo affrontare con serietà questi argomenti, visto che poi

considero corretto, perché c'è bisogno di avere un'agenzia che crei *software* e *hardware,* ma che sia un punto di riferimento sia per il pubblico sia per il privato. Da questo punto di vista, il tipo di strutturazione che si dà a quest'agenzia mi convince molto, perché i molto, perché i problemi che erano sorti in una prima ipotesi nel Governo precedente e che sembravano non delineare bene i confini fra le Agenzie di *intelligence* e il ruolo di questa adesso

Questo è un tema cruciale per il futuro di qualsiasi Paese e per la sicurezza dell'economia, dello sviluppo, della crescita, ma anche della vita, come ha dimostrato la storia di quella povera signora tedesca. tedesca. Il cambiamento culturale che dobbiamo fare è fondamentale, perché, quando riceviamo un attacco, siamo già in ritardo.

che è l'inizio di una *road map* che deve prevedere la messa in sicurezza della pubblica amministrazione, l'educazione e la formazione dalla scuola è importante che si capiscano i rischi), gli investimenti, le assunzioni, le collaborazioni internazionali e anche l'adeguamento del quadro politico giuridico nazionale e internazionale. Il tema, infatti, sarà anche come si perseguono questi reati quando gli *hacker* sono stranieri non identificati, che però producono danni terrificanti all'economia o alla sicurezza di una Nazione. Abbiamo quindi davanti un percorso che comincia, ma certo non finisce con oggi; oggi però decidiamo qualcosa che è necessario e importante.

I fatti di queste ultime ore ci dicono che siamo arrivati in ritardo e che le polemiche nei confronti dell'ex presidente Conte erano pretestuose, perché era stato proprio lui a proporre un ragionamento serio su queste questioni. I fatti di queste ore ci dicono anche che dobbiamo rapidamente recuperare il tempo perso e rendere operativa l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Colleghe e colleghi, era già scritto purtroppo. Sono andato a rileggere le pagine di un libro, «Guerra senza limiti. L'arte della guerra asimmetrica fra terrorismo e globalizzazione», scritto sul finire degli anni Novanta da due colonnelli cinesi commissari politici dell'esercito cinese - la prefazione in italiano è del generale Fabio Mini - che avevano previsto attentati come quello alle Torri Gemelle, analizzando i nuovi scenari bellici in chiave di guerre asimmetriche e spiegando il terrorismo e le sue tecniche; le guerre asimmetriche vengono condotte attraverso la manipolazione dei *media*, le turbative dei mercati azionari, la diffusione di virus informatici, le azioni di pirateria sul *web* e la manipolazione del voto. Oggi prendiamo drammaticamente atto di questi nuovi scenari bellici. Capisco il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, quando afferma che l'attacco informatico nel sistema virtuale gestito da LAZIOcrea è un atto di terrorismo. Sì, è terrorismo, anche se i pirati informatici hanno chiesto il riscatto. Pensiamo agli effetti provocati, al blocco totale delle prenotazioni vaccinali e alle visite in ospedale nelle ASL che sono ferme; per la gestione degli appalti e del pagamento del bollo per i veicoli e delle tasse regionali. Se fino a qualche tempo fa gli *hacker* rubavano segreti aziendali per ricatto, estorsione o per rivenderli ai concorrenti, quello che è certo è che la digitalizzazione ha avuto una forte accelerazione con la pandemia e quindi oggi mettere in sicurezza i dati è assolutamente fondamentale per la sicurezza del Paese. Sotto attacco possono finire tutti gli enti, quelli istituzionali innanzitutto, aziende pubbliche e private. Dopo l'attacco *hacker* alla Regione Lazio, infatti, l'antiterrorismo teme che altri siti istituzionali possano essere violati. Nel 2020 - ci dicono gli esperti - ci sono stati 156 episodi di *cybercrime* o di cyberspionaggio al mese; quest'anno attacchi informatici hanno bloccato ospedali, gasdotti e impianti di purificazione dell'acqua in città. Quanto sta accadendo nel Lazio è la dimostrazione plastica di quanto sia importante che lo Stato appronti le migliori soluzioni possibili per scongiurare il verificarsi di episodi simili. La vulnerabilità dei sistemi informatici è un rischio che la pubblica amministrazione non può permettersi di correre, perché la assoggetterebbe al pericolo del rallentamento, quando non di una vera e propria paralisi dell'azione amministrativa, inoltre può essere fonte di danni rilevantissimi sul fronte della violazione di dati personali e della loro divulgazione o mercificazione. L'emergenza Covid ha poi dimostrato che un uso maggiore degli strumenti informatici e delle connessioni in rete amplifica le occasioni di attacco. Come si legge nella relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2020, la pandemia è stato un evento determinante anche in termini di impatto sulla società, sulle tecnologie in uso alla popolazione, sulla digitalizzazione di attività e servizi, nonché sul conseguente ampliarsi della superficie di rischio cibernetico per l'individuo e per l'intero sistema Paese. Hanno quindi acquisito maggiore attualità e concretezza le minacce alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, nonché alla continuità degli approvvigionamenti. Nel complesso, si è evidenziato come gli attori ostili abbiano sfruttato nel periodo pandemico il massiccio ricorso al lavoro agile e la conseguente accessibilità da Internet di risorse digitali di Ministeri e aziende di profilo strategico e infrastrutture critiche, divenuti ancor più bersaglio di campagne ostili. Colleghe e colleghi, la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 13 luglio 2021. In particolare, in tale ambito, la *cybersecurity* è uno dei sette investimenti della digitalizzazione digitalizzazione della pubblica amministrazione. Avete sentito la collega Pinotti ricordare le dichiarazioni del ministro Colao: il 95 per cento dei *server* della pubblica amministrazione non è sicuro. È vero, bisogna correre. Abbiamo bisogno di sviluppare in tempi brevi, idonei e sempre più serrati meccanismi di tutela. Altri Paesi hanno investito nella sicurezza informatica da anni, come la Francia e la Germania. Appare quindi urgente intervenire rinforzando il sistema di difesa contro questo genere di reati, che possono rivelarsi particolarmente insidiosi e creare danni ingenti. L'istituzione dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, del Comitato interministeriale per la cybersicurezza e, nell'ambito di quest'ultimo, del nucleo per la cybersicurezza sembra essere un passo in avanti nell'ammodernamento del sistema di sicurezza nazionale. Per questo motivo, dichiaro il voto a favore delle senatrici e dei senatori di Liberi

Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento e ovviamente aggiungiamo anche noi alcune considerazioni rispetto alla vicenda. In un libro pubblicato in occasione dei quarant'anni dall'insediamento di Ronald Reagan alla Casa Bianca, una biografia del Presidente americano scritta dal giornalista Gennaro Sangiuliano, uno dei capitoli finali parla della vittoria nella Terza guerra mondiale, che è stata attribuita a Reagan. Qualcuno si potrebbe chiedere quale sia stata questa Terza guerra mondiale. Fu una guerra. All'epoca c'erano ancora i blocchi classici che facevano capo agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica, che era ancora tale. la frontiera tecnologica era lo scudo spaziale

e che oggi ha portato, pur con mille problemi nel mondo, a un diverso assetto. Oggi c'è una guerra in corso ed è stata già descritta da molti colleghi: è la guerra delle tecnologie, gli attacchi del *cybercrime,* che sono in corso. Non mi voglio agganciare all'attualità, perché sinceramente l'attacco che c'è stato nel Lazio è grave ma non è il primo; voglio capire, però, perché mi ricordo che anche l'INPS qualche tempo fa se la prese con gli *hacker*

Ho letto oggi notizie di dipendenti che avrebbero avuto accesso a siti pornografici che contenevano virus; non lo so. Quando avremo l'Agenzia, questa riuscirà anche a distinguere la dabbenaggine tecnologica dagli attacchi, quindi non esprimo giudizi. nazionale per la cybersicurezza, perché riteniamo che oggi la difesa delle frontiere digitali sia importante tanto quanto quella delle frontiere fisiche, quindi riteniamo che sia assolutamente necessario attrezzarsi. Sulle frontiere fisiche invitiamo anche il Governo a una maggiore attenzione: non vorrei che essersi concentrati sull'Agenzia per la *cybersecurity* abbia fatto un po' mollare la guardia sui confini fisici, ma questa è un'altra storia. allora che sia assolutamente necessario dotarci di questo strumento. Oggi gli interventi dei colleghi del Gruppo Forza Italia non hanno sottaciuto alcune criticità.

banche dati e attacchi sono possibili in tutti gli ambiti. L'attacco di cui si parla sta impedendo di avere il *green* *pass* o di prenotare i vaccini; non è stata attaccata una struttura di difesa, perché i dati sono ovunque. Oggi, a volte, esistiamo più nella percezione digitale che non in quella fisica. Sembra un paradosso, ma è così; quindi, è assolutamente necessario agire in questa direzione. Oggi il mondo può essere bloccato, perché, essendo connesso, basta bloccare la connessione per paralizzarlo. Ringrazio i membri del Governo presenti; forse gli impegni non hanno consentito al membro del Governo che è Autorità delegata di assistere a questo dibattito, ma sarebbe stato utile.

e si è fatto tardi rispetto alla storia. Non ripercorro qui la cronistoria, come molti hanno fatto, sulle direttive europee, sulle sollecitazioni internazionali e sulle emergenze di ogni genere e tipo che rendono necessaria quest'Autorità,

Ci auguriamo che quest'Autorità e questa struttura funzionino bene. Non sarà facile, perché si deve raccordare con l'attività ordinaria dei servizi di sicurezza, che restano competenti per tutte le loro funzioni, che svolgono egregiamente, con le altre autorità militari, di difesa, e con tutte le altre autorità ministeriali. Nel nucleo molti sono rappresentati e diranno la loro, ma alcuni sono assenti, quindi è un mondo complesso. Si è anche discusso del trattamento del personale. Noi, che saremo la casta per eccellenza siamo circondati da caste. Io pure avrei preferito che, invece di dare il trattamento del personale della Banca d'Italia

occorre anche un trattamento economico adeguato. Si agisce in ritardo e bisogna intervenire: servono intelligenze, come poc'anzi anche il senatore Aimi ricordava nel suo intervento; non si mette in piedi un ufficio con 300 persone scelte a caso, ma serviranno competenze, perché le attività della criminalità

in tutti i vari comparti questa consapevolezza e questa necessità di difesa dei confini tecnologici, quindi guarderemo anche noi con un voto favorevole, dato con sincera predisposizione, come funzionerà questa cosa.

tecnologica, nella modernizzazione delle reti e quindi anche nella *cybersecurity*. Dobbiamo quindi assolutamente metterci in scia, utilizzare questi fondi e rendere il Paese più sicuro,

si distraggono di fronte al Grande fratello quotidiano che si compra la nostra vita. Basta ordinare una pizza con *delivery* e hanno tutto della nostra vita e dei nostri dati. Non parliamo di Amazon,

*privacy*. Non possiamo rinunciare a prenotare un cibo con il telefonino o a fare acquisti a distanza, tuttavia credo che anche qui un po' come la storia del *green pass* o dei vaccini: ci si preoccupa di alcune cose, ma si trascurano forme di appropriazione della nostra vita e della nostra identità

quindi a favore, sperando che questa struttura ci aiuti a difendere la libertà e la sicurezza del Paese, una difesa su frontiere moderne e innovative, ma sappiamo che c'è ancora molto da fare per la nostra libertà e la nostra sicurezza.

di questi tempi molti Paesi sono sempre più bersaglio di attacchi *cyber*. L'Italia non ne è esente, anzi il nostro Paese è tra i più vulnerabili e dunque tra i più colpiti da minacce informatiche insidiose, sempre più numerose e diversificate, talune messe in atto da gruppi criminali, che possono chiedere un riscatto oppure vendere sul mercato le informazioni sottratte, ed altre messe in atto da attori statuali, con lo scopo di rubare informazioni sensibili, ad esempio su terapie, ricerche o brevetti. I cyberattacchi sono in forte aumento anche a seguito della transizione digitale, del forte sviluppo e implementazione dell'intelligenza artificiale, dell'Internet of things, della tecnologia 5G e del forte aumento del traffico in Rete causato dal Covid, che ha costretto milioni di persone, lavoratori e studenti a lavorare da remoto e a studiare con la didattica a distanza (DAD), determinando un'esplosione degli attacchi informatici. La cybersicurezza è diventata così una priorità assoluta per lo Stato, le istituzioni, le aziende e i privati, che devono assolutamente ridurre il loro grado di vulnerabilità. Ricordo quando il Copasir, da sempre attento ai temi della sicurezza *cyber* e delle sue implicazioni sulla sicurezza nazionale, con la relazione sul 5G rilasciata al Parlamento nel dicembre 2019 sottolineò i forti rischi con particolare riferimento all'impiego di apparecchiature e tecnologie cinesi nelle infrastrutture italiane. *(Applausi)*. Fu un appello che per diversi mesi è rimasto inascoltato dal Governo precedente. Non è un caso quindi che la sicurezza cibernetica costituisca uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. In coerenza con il PNRR, però con diversi anni di ritardo rispetto a Germania e Francia, che hanno già operativa da tempo una struttura consolidata che opera per difendere i rispettivi Paesi dalle minacce cibernetiche, accogliamo con favore questo decreto-legge, che definisce l'architettura nazionale di cybersicurezza e fa nascere anche in Italia un'Agenzia *cyber* nazionale, che determina un passaggio cruciale per la sicurezza nazionale nel nostro Paese. Tale razionalizzazione porta ad avere da ventitré soggetti competenti, ma dispersivi, che dialogavano su questa materia, ad un unico soggetto pubblico, che sarà l'interlocutore in Europa e nello scenario internazionale sui temi *cyber.* Sarà un'Agenzia strutturata, dotata inizialmente di trecento unità di personale, che entro il 2027 potrebbero arrivare addirittura a ottocento. Saranno figure di alta professionalità, oggetto di continua formazione, in grado di raggiungere i livelli di produzione *hardware* e *software* necessari per dotare il nostro Paese di autonomia tecnologica e renderci competitivi in campo internazionale. Il provvedimento ci arriva blindato dalla Camera, dov'è stato oggetto di non molte modifiche, ma alcune comunque importanti che hanno visto il contributo decisivo della Lega, come quello che ha eliminato ambiguità e rischi di sovrapposizione delle competenze della nuova Agenzia con quelle delle nostre Forze di polizia, che continueranno le indagini ...come quelle della nostra difesa, che continuerà a contrastare gli attacchi alle infrastrutture militari con la cyberdifesa e come quelle della nostra *intelligence*, il DIS e le Agenzie AISE e AISI, sulla raccolta delle informazioni. esame è un provvedimento importante, che si distingue nettamente dal pessimo e opaco progetto che il Governo Conte-*bis* lo scorso novembre stava inopportunamente proponendo nel disegno di legge di bilancio 2021 e che ipotizzava la costituzione di una fondazione sulla cybersicurezza, incardinata nel perimetro del DIS, ma con la previsione di uno statuto di cui non vi era contezza di contenuto. vi sarà un'accelerazione del cambio di paradigma, che punta alla resilienza, alla prevenzione del rischio e della minaccia, con lo sviluppo di strumenti di *safety*, che si aggiungono agli strumenti di repressione e contenimento, cosiddetti di *security*, che vedrà da un lato sempre più investimenti sulle competenze digitali dall'altro, vedrà lo Stato proteggere da attacchi informatici i sistemi pubblici, vigilando così sull'erogazione di servizi fondamentali per i cittadini. Oggi occorre dunque accelerare sulla costituzione e sulla operatività dell'Agenzia, abbiamo oltre il 90 per cento dei *server* della pubblica amministrazione non in condizioni di sicurezza, per non dire che alcuni sono dei colabrodo e quindi non siamo sicuri. il violento, invasivo e criminoso attacco *hacker* proveniente dall'estero, forse dalla Germania, ma con probabile triangolazione, che dalla scorsa domenica notte ha colpito e infettato i *server* del CED della Regione Lazio, paralizzando anche il portale "Salute Lazio" e la rete vaccinale, bloccando le prenotazioni dei cittadini, dimostra quanto ormai sia indifferibile rendere operative le difese *cyber*, anche perché i danni sono molto gravi. La Regione è ancora in ostaggio e forse lo sarà per giorni e sulla vicenda stanno indagando i pubblici Forse è scongiurato che gli *hacker* abbiano avuto accesso alla storia sanitaria di milioni di cittadini laziali, ma comunque pare certo che i dati sono stati criptati e resi inservibili, compreso il *backup*. Purtroppo quello del Lazio non è il primo attacco che accerta la vulnerabilità del settore sanitario, che è uno dei bersagli più delicati in tempo di pandemia. Ricordo come nel marzo dello scorso anno, in pieno *lockdown*, *hacker* avevano preso di mira il "San Raffaele" di Milano e poi, in aprile, l'ospedale "Spallanzani" di Roma, senza contare gli attacchi non resi pubblici. un'ultima considerazione, prima delle conclusioni, con riferimento al Copasir, da cui - lo rammento - io e il collega deputato Volpi, allora Presidente, ci siamo dimessi, invitando tutte le forze politiche a fare altrettanto, per ragionare

nella convinzione che occorresse, allora come anche oggi, procedere necessariamente ad una attualizzazione della stessa legge disciplinante il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

la modalità di azione dell'Autorità delegata, che prima aveva esclusivamente un rapporto con le Agenzie del comparto di *intelligence* o comunque con il sistema della sicurezza luogo, perché è cambiato anche il momento storico e tecnologico, da quando la legge è stata approvata. Dunque la Lega ritiene che un tagliando alla legge n. 124 sia non più differibile la garanzia della presenza paritaria dei componenti del Copasir, che sarebbe opportuno diventasse proporzionale rispetto alle forze di maggioranza e minoranza di Governo, non valga solo per l'opposizione, ma anche per la stessa maggioranza, che deve in futuro potersi trovare nella condizione di poter scegliere il Presidente in votazione segreta, tra più candidati. confermando il voto favorevole della Lega su questo provvedimento e ovviamente augurando buon lavoro a tutti i soggetti che saranno protagonisti nella futura istituenda Agenzia per la cybersicurezza

Presidente, nell'affrontare questo provvedimento circa le disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, la definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale non si può omettere come oggi si colmi un ritardo; al tempo stesso, il provvedimento rappresenta anche un tassello ulteriore nella più generale necessità di sviluppare in tempi brevi idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela cibernetica. Per anni l'Europa ci chiedeva un interlocutore certo, definito e unitario sui temi della cybersicurezza, ma il nostro Paese si presentava con 23 soggetti competenti che interloquivano su questa materia. È stata fatta una scelta di resilienza cibernetica (dunque strutture, professionalità e formazione), necessaria a dotare il Paese di un'autonomia tecnologica che consenta di raggiungere livelli di produzione *hardware* e *software* che ci rendano che ci rendano competitivi nello scenario internazionale. In capo c'è un soggetto pubblico, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che dialoga con pubbliche amministrazioni e soggetti privati, con il compito non solo di definire *standard* di sicurezza applicata ai vari contesti, ma anche di coordinare eventuali sovrapposizioni con il mondo militare e dell'*intelligence*. L'Italia non solo non può permettersi di rinunciare al progresso digitale, evitando di utilizzare tecnologie a causa di potenziali minacce introdotte, ma è anzi chiamata a usarle e gestirle al meglio, nella piena consapevolezza dei rischi, per poterne godere i benefici. I rischi per la sicurezza informatica impattano anche sul progresso economico e sociale di un Paese. La creazione di una struttura *ad hoc*, con la direzione nelle mani dell'attore pubblico, è ormai improcrastinabile. Il provvedimento che ci accingiamo a votare è il compimento di un processo di definizione e ricomposizione di funzioni e compiti attinenti al settore della cybersicurezza, quale ambito delicato e al contempo ancora troppo vulnerabile. Nel 2019, come evidenziato nel corso delle audizioni sul decreto-legge in esame alla Camera dei deputati, sono aumentati del 246 per cento gli attacchi alle nostre infrastrutture critiche e ancor più il processo di transizione digitale e il massiccio aumento del traffico in rete dopo la prima ondata di Covid hanno costretto a milioni di persone e lavoratori del mondo, portando con sé inevitabilmente un'esplosione degli attacchi informatici. Al centro delle recenti cronache giornalistiche c'è anche quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi ai sistemi informatici della Regione Lazio, in particolare al centro di elaborazione dati, il sistema che gestisce l'intera infrastruttura informatica regionale. Appena ci si è accorti del problema, per evitare il proliferare dell'attacco e la possibile sottrazioni di dati, i tecnici della Regione hanno disattivato il sistema, di fatto bloccando tutti i servizi informatici regionali, il più importante dei quali in questo momento riguarda la gestione della campagna vaccinale. C'è un brusio un po' troppo forte. Lasciamo intervenire con più tranquillità il collega, grazie. Tuttavia, come inevitabile conseguenza, da domenica il sito della Regione Lazio e tutti i siti legati ai servizi informatici regionali sono irraggiungibili. La piattaforma regionale per la prenotazione degli appuntamenti delle vaccinazioni è bloccata; questo significa, in altri termini, che dal 13 agosto non sarà possibile prenotare le vaccinazioni. Se non si riattiva il servizio, al contempo è impossibile prenotare visite specialistiche, sono interrotti gli *screening* programmati, i cittadini e le imprese laziali non possono ottenere diverse autorizzazioni sanitarie ed edilizie, proprio perché sono bloccati anche tutti i servizi informatici non sanitari che di solito fanno riferimento alla Regione Lazio. Questo incidente fa perciò capire quanto la superficie di vulnerabilità sia cresciuta e quanto questa materia sia davvero importante e fondamentale. Dotare il nostro Paese di una nuova normativa che introduca contromisure volte a potenziare le nostre difese informatiche e prevenire attacchi ad infrastrutture di interesse nazionale è più che mai prioritario.

Tale esigenza è infatti aumentata negli ultimi anni, anche alla luce delle misure volte a garantire infrastrutture *cloud* sicure e centri di elaborazione dati con elevati *standard* di qualità, nella direzione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni. Inoltre, la sicurezza cibernetica costituisce uno degli strumenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 31 luglio 2021. In tale ambito la *cybersecurity* è uno dei sette investimenti della digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione», compresa nella missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo». parte, la difesa e la sicurezza nazionale e cibernetica pervadono e influenzano anche lo sviluppo economico, dall'altra parte la *privacy* di milioni di persone e la sanità, come nel caso specifico della Regione Lazio, della purtroppo non esclusa doppia estorsione (criptazione, da un lato, e sottrazione dei dati, dall'altro), devono spingerci ad approvare oggi in Assemblea un provvedimento che vada in questa direzione e che, tra l'altro, istituisce un'apposita Agenzia, che svolgerà il ruolo di Autorità nazionale per la cybersicurezza, al fine di assicurare un'azione unitaria e coordinata in tale settore, per proseguire e completare la strada intrapresa con il cosiddetto perimetro di sicurezza cibernetica. Per tali motivi, il MoVimento 5 Stelle voterà favorevolmente su questo provvedimento.

ieri si sono svolti a Mantova i funerali del professor Giuseppe De Donno, ex primario di pneumologia dell'ospedale di Mantova, noto per essere stato il pioniere della terapia sperimentale anti-Covid a base della trasfusione di plasma iperimmune. Qualche mese fa, su richiesta del MoVimento 5 Stelle, avevamo invitato il professore in Commissione sanità al Senato per presentare i risultati dei suoi studi. Ricordo ancora con quale fierezza il professore, in quella sede, rivendicasse il ruolo avuto dalla sua *equipe* nella gestione della prima fase della lotta a questa pandemia. Ricordo anche, però, il dibattito che nacque in quel periodo sulla validità o meno di questa terapia, scatenando una guerra mediatica e politica, che metteva in contrapposizione i vaccini - che, in realtà, sono strumenti di prevenzione - con le terapie, soprattutto domiciliari, che invece sono strumenti di cura. In questi mesi la scienza, attraverso i nostri medici e i nostri ricercatori, ha dato il meglio di sé, facendo passi da gigante per comprendere questa nuova malattia e combatterla nel modo più efficace. Dall'inizio di questa pandemia ad oggi è cambiato totalmente l'approccio ai pazienti Covid: abbiamo imparato che bisogna intervenire quanto prima e le cure precoci con plasma di soggetti immuni e con anticorpi monoclonali hanno certamente rappresentato un'arma efficace. efficace. Grazie alla nostra esperienza, gli altri Paesi europei e mondiali hanno avuto più armi per curare i propri malati. Il professor De Donno ha certamente contribuito allo sviluppo di queste conoscenze. Era un ottimo medico, stimato dai colleghi, dai suoi pazienti, una mente brillante, un uomo riservato e schietto, certamente non avvezzo al clamore mediatico che gli è stato riservato, né credo avesse mai voluto diventare argomento di scontro politico. Al professor De Donno dico grazie per il suo contributo, per aver vissuto da vicino il dramma del Covid e anche la rinascita di chi, grazie alla sua terapia, ce la faceva. Resta nel nostro cuore la tristezza per una vita che si spegne e l'amarezza per aver dedicato fino ad oggi poca attenzione alle terapie domiciliari. Da parte mia, dei miei colleghi di Commissione e di tutto il mio Gruppo, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia ai suoi colleghi. Questa morte è un dolore immenso per noi ed anche una grande sconfitta per non aver saputo proteggere e tutelare coloro che chiamiamo eroi, ma che abbiamo lasciato soli nei reparti a gestire carichi di lavoro non tollerabili e senza supporto psicologico.

in cui persero la vita 85 innocenti e oltre 200 furono i feriti. Dopo quarantuno lunghi anni si conosce solo un pezzo di verità di quella orrenda strage terroristica, che è la più grave della storia repubblicana. Sono stati condannati in via definitiva gli esecutori materiali, individuati nei terroristi neofascisti Valerio Fioravanti, Luigi Ciavardini e Francesca Mambro, ma è in corso un ultimo processo che vede imputato Paolo Bellini, che è un soggetto che è stato ripreso da un turista sul luogo della strage pochi minuti prima. Sono stati poi condannati anche i depistatori di Stato, tra cui alcuni dirigenti infedeli del Sismi, l'allora servizio segreto militare, come il generale Musumeci e il colonnello Belmonte, oltre al faccendiere Pazienza e al gran maestro della loggia P2 Licio Gelli, che tutti insieme cercarono di proteggere gli esecutori materiali e di soffocare in tal modo la verità. Dopo quarantuno anni, Presidente, i mandanti non sono stati ancora individuati e condannati, anche se alcuni documenti, che recentemente sono tornati magicamente alla luce, indirizzano le indagini verso Licio Gelli e Umberto Ortolani e gli ambienti della P2 che avrebbero corrisposto ingenti somme ai terroristi qualche giorno prima della strage. Queste indagini si rivolgono anche verso Federico Umberto D'Amato, che era a capo dell'Ufficio affari riservati del Ministero dell'interno, e a Mario Tedeschi, giornalista della rivista Purtroppo sono ancora sconosciuti gli ispiratori politici di quell'attacco al cuore dello Stato e alla nostra democrazia, anche se non è difficile immaginare a quale ambito appartenessero. Valerio Fioravanti, ex baby attore, ex militante del Movimento Sociale, ex terrorista dei NAR, esecutore e/o mandante di otto omicidi, tra cui poliziotti e magistrati, esecutore - come dicevo per tutto questo ha scontato solo diciotto anni di carcere e circa otto in regime di semilibertà. Dal 2009 è libero. Durante la detenzione, anzi più esattamente durante le udienze dei vari processi in cui era imputato, ha avuto il tempo di fare un figlio con la sua compagna, anche lei terrorista, neofascista e coesecutrice della strage. Tra un omicidio e l'altro, tra una rapina e l'altra, assaltava cinema che proiettano i film di Pier Paolo Pasolini insieme ai suoi camerati, oppure le radio private che si interessavano di politica e facevano parlare militanti sindacali o militanti femministe. Smettere di battersi per la verità storica e processuale e pensare che ormai è passato troppo tempo per accettarla sarebbe fare un favore ai fascisti come Fioravanti, Mambro, Ciavardini e ai loro mandanti e darla vinta a chi voleva uccidere, nel terrore, la nostra democrazia e la nostra libertà.

ho apprezzato l'annuncio che proprio ieri, a Bologna, ha dato il ministro della giustizia Cartabia, dicendo che alcuni documenti riguardanti vicende della P2 e altri accadimenti di quegli anni saranno desecretati.

di cui facevo parte insieme al senatore Giovanardi e altri colleghi. Chiedemmo la desecretazione di una serie di documenti che abbiamo letto nei vincoli di riservatezza che la Commissione di inchiesta ha

Le vicende di quella tragica estate videro prima la vicenda di Ustica, mai realmente chiarita fino in fondo, e poi la vicenda di Bologna, per la quale c'è una verità giudiziaria accertata.

il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha parlato di una mistificazione su queste vicende. Sì, c'è una mistificazione, ma a mio avviso la si scopre guardando quelle carte. Il giornalista Grignetti, su «La Stampa» le ha pubblicate anni fa, quindi è il segreto di Pulcinella. I rapporti che venivano dal Medio Oriente in quegli anni fanno capire chiaramente la matrice della vicenda di Ustica e della strage di Bologna. Quei documenti smentiscono in maniera totale le verità giudiziarie accertate, sulle quali si costruiscono leggende che anche prima ho sentito riecheggiare in quest'Aula. Insisto affinché vengano desecretati quegli atti rapporti del colonnello Giovannone dal Libano, che dicono chi ha fatto Ustica e chi la strage di Bologna, smentendo sentenze basate su fatti non reali. Infatti, i fatti reali e quei rapporti riservati dicono un'altra verità, che però qualcuno non vuole ascoltare per continuare a fare le leggende, come abbiamo sentito anche questa sera